*relatore*. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, abbiamo oggi in esame il disegno di legge che il Governo ha presentato per la sospensione di tre decreti attuativi della riforma dell'ordinamento giudiziario predisposta dal Governo e approvata dal Senato nella precedente legislatura. Com'è noto, tale riforma dell'ordinamento giudiziario, essendo stata realizzata con lo strumento della legge delega, prevedeva molteplici decreti delegati. Alcuni di essi, tre per l'esattezza, che al momento della predisposizione e della presentazione del disegno di legge da parte del Governo non erano ancora entrati in vigore, concernono aspetti molto rilevanti della disciplina dell'ordinamento giudiziario. Il primo di essi tratta le materie dell'accesso alla magistratura, della progressione in carriera, della formazione professionale, il secondo riguarda la nuova organizzazione del sistema delle procure della Repubblica; il terzo concerne l'ordinamento disciplinare. Come ricordavo, al momento della presentazione del disegno di legge quei decreti legislativi non erano ancora entrati in vigore.

che pure si era ipotizzato, della decretazione d'urgenza; non si è ritenuto, giustamente, di inserire la sospensione di questi provvedimenti, come pure sarebbe stato tecnicamente possibile, in uno dei provvedimenti che il Governo ha assunto per il rinvio di termini in altri campi. Si è ritenuto di seguire la via dell'ordinario disegno di legge e così si è fatto, dapprima nella sede della Commissione giustizia, dove c'è stato un serrato e ampio confronto (e devo dare atto a tutti i colleghi della Commissione, della maggioranza e dell'opposizione,

in questo ramo del Parlamento -, l'ordinaria procedura parlamentare, come è giusto, senza contingentamento dei tempi. Pur nella serenità del confronto, è evidente che sono emerse, tanto in sede di Commissione come nella discussione generale che abbiamo svolto, posizioni che hanno visto contrapposte la maggioranza e l'opposizione. In sé non ci sarebbe da stupirsi di questo: l'attuale opposizione difende una legge che ha fortemente voluto nella passata legislatura, la maggioranza adempie, con questo strumento, a un impegno assunto nel suo programma elettorale, quello di modificare profondamente la disciplina dell'ordinamento giudiziario, così come prevista nei decreti delegati. Perché si è seguita questa strada? Sono risuonati anche nel corso della discussione generale argomenti ai quali intendo brevemente replicare: non si tratta, come è stato detto, di un cedimento alle pressioni dell'Associazione nazionale magistrati o della magistratura in quanto tale. Non si tratta di questo, perché la necessità di un profondo cambiamento dell'ordinamento giudiziario, eventualmente anche con la sospensione dei relativi decreti delegati, era stata presentata davanti ai cittadini nel programma dell'Unione. Quindi non c'è - mi rivolgo al collega Caruso - alcuna cambiale sottobanco da pagare, ma c'è un impegno assunto davanti agli elettori. Se una cambiale, che viene

Perché, ci si potrebbe domandare, questa nostra scelta? Vorrei ricordare innanzitutto che il Governo non ha proposto l'abrogazione di quei decreti delegati, ma la loro sospensione. Non ha proposto l'abrogazione perché, come ha ricordato il ministro Mastella nel suo intervento prima della discussione generale, noi riteniamo che ci siano dei cambiamenti profondi da apportare nell'ordinamento giudiziario preesistente la riforma Castelli. È giusto che la definizione di questa nuova disciplina che si deve introdurre avvenga con il concorso dell'opposizione, da ricercare - lo diceva bene ieri il senatore Manzione - nell'Aula parlamentare e non in comitati ristretti esterni al Parlamento, che pure sono stati ventilati,

Vorrei richiamare solo che le ragioni per cui chiediamo le modifiche di questo testo sono legate a quanto ha detto il senatore D'Ambrosio nel suo intervento: l'ordinamento giudiziario non è materia che riguarda la professione dei magistrati, ma è materia che deve essere affrontata innanzitutto dal punto di vista dei diritti dei cittadini. cittadini. Il tema dell'autonomia e dell'indipendenza, così come quello della responsabilità del magistrato, deve quindi essere affrontato sul versante del diritto del cittadino ad una magistratura autonoma, indipendente e responsabile. Noi riteniamo che nell'impianto dell'ordinamento giudiziario, così come approvato dalla precedente maggioranza, non ci sia questa attenzione alla centralità del diritto del cittadino. Se volessi fare una considerazione al riguardo, mi pare che trapeli una certa nostalgia per una magistratura del passato, che pure abbiamo conosciuto, una magistratura gerarchizzata nella quale la Corte di cassazione funzionava effettivamente come strumento di controllo e di selezione della magistratura e l'organizzazione gerarchica delle procure funzionava come modo per limitare o controllare l'esercizio dell'azione penale: la magistratura degli anni Cinquanta, in breve, che aveva una chiara connotazione sociale, conservatrice e talvolta francamente reazionaria. Ma oggi la magistratura, a tutti i suoi livelli, non è più così e anche la svalutazione del ruolo del giudice di primo grado (che è il giudice di frontiera, il magistrato che più deve affrontare i temi dei diritti dei cittadini) è a mio avviso profondamente sbagliata. Ciò vuol dire chiusura totale al confronto? Credo di no. Ad esempio, il senatore Mantovano ha svolto sull'articolo 3 di questo provvedimento considerazioni critiche che io in larga misura condivido, come già ho avuto modo di dire in Commissione e al riguardo avremo occasione di pronunciarci in sede di esame di tale articolo. Il senatore Manzione ieri ha svolto un intervento coerente - ma forse il senatore Zanda non l'ha seguito,

ha svolto considerazioni per altro coerenti con la posizione sostenuta in Commissione e, devo dire, avvalorate anche dall'intervento svolto l'altro giorno Il Ministro ci ha delineato possibili linee di una proposta del Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, che dovremo affrontare in sede - come è nostro impegno fare - appena completata la sospensione (se questa verrà approvata dal Parlamento). Naturalmente, il disegno di legge ancora non c'è, ma le linee sono state chiaramente indicate. Ed effettivamente l'impostazione del Governo, che poi spetterà al Parlamento esaminare, mentre mi pare sostanzialmente alternativa cosiddetti decreti Castelli (quelli riguardanti accesso, funzioni e così via), è emendativa - ragionevolmente - degli altri due. Per le procure, non si può tornare alla situazione preesistente, anche se è sbagliato l'impianto gerarchico del sistema attuale; in merito al sistema disciplinare, una volta accolto - come ha fatto il Governo - il principio dell'obbligatorietà, i problemi mi pare che siano due, relativamente semplici da affrontare: individuare un meccanismo di filtro, per evitare che l'obbligatorietà dell'azione disciplinare comporti una dispersione dei tempi, e rivedere alcune fattispecie della tipicità.

dal Governo, con una precisazione che mi permetto di fare in Aula al Ministro (se il sottosegretario Pinza gli consente di ascoltare). Ho sentito dal senatore Ciccanti un'osservazione critica su una frase del Ministro, che credo sia stata una *boutade*, quando ha parlato di titoli preferenziali per parlamentari, senatori, consiglieri comunali per l'accesso in magistratura. È evidente che non possiamo immaginare un ordinamento giudiziario in cui vi siano norme di preferenza per il ceto politico: sconsiglierei, quindi, di seguire tale strada, anche persino in termini di presentazione di un disegno di legge, perché condivido il rilievo critico espresso dal senatore Ciccanti. Voglio concludere auspicando un clima disteso nel confronto parlamentare, come ha invitato a fare il Presidente della Repubblica nell'indirizzo di saluto rivolto ai componenti del Consiglio superiore della magistratura l'8 giugno 2006, qui richiamato dagli equilibrati interventi dei colleghi dell'UDC. È un discorso che vale per noi in Parlamento, per le categorie professionali e per la stessa magistratura. Ci ha detto il Capo dello Stato: «Occorre superare le tensioni fra politica e giustizia, inevitabilmente destinate a turbare lo svolgimento di una così alta funzione costituzionale. Il recupero di toni che non siano di pura contrapposizione agevola la ricerca di punti di convergenza. Il dialogo è premessa indispensabile per restituire funzionalità al sistema giustizia». Questa è organizzazione fondamentale, come dicevo all'inizio, per tutelare i diritti dei cittadini e, soprattutto, dei cittadini più deboli nella società. Sono infatti i cittadini più deboli che hanno il diritto a che il Parlamento eserciti la sua funzione pensando a loro, hanno diritto a una magistratura certamente responsabile, ma anche autonoma e indipendente, perché se tale non è dipenderà da qualcuno e non sarà certamente dai cittadini comuni, ma piuttosto da potentati politici, economici o finanziari. Con tali considerazioni, ritengo che questo provvedimento sia meritevole di approvazione ed auspico che il confronto parlamentare si svolga, nella contrapposizione fisiologica propria di una democrazia parlamentare, tenendo conto dell'esigenza di una convergenza, mai come in questa materia, alla ricerca del bene comune.

innanzitutto mi sia consentito ringraziare i colleghi che da vari appezzamenti politici e di territorio

Non ho inteso proporre, e lo dico anche all'amico senatore Manzione, alcuna controriforma. Mi pare che l'impianto di per sé, le linee di convergenza che ho tentato di tracciare, lo stesso fatto che alcuni decreti da me sostenuti, precedentemente legittimati sul piano parlamentare dal ministro Castelli, siano stati recepiti e portati a compimento e all'efficacia operativa, dimostrino che non c'era la voglia matta di operare in controtendenza, con una visione antagonistica, con uno sforzo pregiudiziale a tutti i costi: assolutamente non è stato così. Però, lo voglio ricordare a me stesso e agli altri, c'è stato uno spartiacque elettorale, esiste un programma al quale ho il dovere di attenermi. Che questo programma consenta di attenersi a quanto è stato scritto, mi pare evidente; che poi ci sia, come c'è sempre stato, e rimane sullo sfondo, dal mio punto di vista, la volontà di dialogare e trovare motivi di convergenza, questo appartiene alla mia cultura e rappresenta anche la linea di fondo lungo la quale si muove questo Governo, per evitare quello che anche il presidente Mancino aveva detto nella sua interlocuzione con il Governo, che vi sia cioè una paralisi nella macchina giudiziaria. Quindi, non c'è il desiderio di favorire lassismi di carriera, di accentuare al tempo stesso la conflittualità tra magistrati e mondo della politica; se vi fosse quindi la possibilità

dando apporto calorico da parte della maggioranza e dell'opposizione, sarei ben felice e lo saremmo tutti quanti. E neppure lo voglio dire a quelli che sono stati più censori dei censori o più soloni rispetto a me, quasi che la mia preferenza fosse di per sé diretta

io abbia tenuto conto degli aspetti che riguardavano le richieste fatte all'Associazione, perché tra le richieste c'erano anche quelle con cui si chiedeva magari di non procedere.

in atto e mi auguro che lo sia. Partendo da questa premessa essenziale, rimane ferma la mia intenzione di predisporre un rigoroso sistema di accesso alla magistratura e un'altrettanto rigorosa progressione in carriera, attraverso severi filtri quadriennali,

in cui oltre alla prioritaria responsabilità del capo ci sia anche quella dei sostituti. Prospetto dunque un passaggio dalla giudicante alla requirente, secondo precise condizioni di specifica professionalità, vietando la permanenza nel medesimo distretto. Ritengo che, tipicizzati gli illeciti disciplinari, per il principio di legalità, l'azione disciplinare non possa che essere obbligatoria, essere obbligatoria, ma con filtri molto severi e molto rigorosi che evitino la crisi della procura generale e della stessa sezione disciplinare. In questa prospettiva rispondo alle obiezioni formulate nel corso del dibattito parlamentare,

se gli aspiranti prima ancora del concorso e poi tutti i magistrati, entro la data fatidica del 28 ottobre di quest'anno, dovranno scegliere tra l'attività giudicante e quella requirente, si verificheranno le seguenti conseguenze, che ho il dovere di sottoporre all'attenzione del Parlamento. La scelta degli aspiranti sarà fatta al buio, senza alcuna consapevolezza di quale lavoro in realtà saranno chiamati a svolgere, senza aver mai sperimentato di persona l'esercizio dell'una o dell'altra funzione e senza aver neppure frequentato un'aula o un ufficio giudiziario. Si spaccherebbe e si spacca in due parti ben distinte la magistratura, abbandonando quel principio di comune cultura della giurisdizione che ogni magistrato deve possedere, pubblico ministero compreso, per non diventare, come si dice a volte, uno spietato «pubblico accusatore». Si determinerebbe e si determina un'enorme confusione nell'assetto concreto degli uffici perché all'opzione deve necessariamente seguire l'esercizio della relativa funzione: insomma, una sorta di terremoto negli uffici, con trasferimenti a catena, scopertura di sedi importanti e asimmetrie distributive al di fuori di ogni politica del personale;

Tale terremoto ricadrà sul funzionamento della macchina giudiziaria e alla fine si depositerà sui cittadini italiani. Come ho già detto, vorrei conservare la distinzione delle funzioni; perciò chi ha fatto il pubblico ministero non potrà di colpo fare il giudice, ma dovrà frequentare un corso qualificante, avere ben precisi pareri del corpo giudiziario e delle rappresentanze dell'avvocatura

Quanto ai concorsi per la progressione in carriera, il vice presidente del CSM, senatore Mancino, ha adombrato, con molto rispetto verso il Parlamento ma con autentica e sofferta preoccupazione, le anomalie tra l'impegno partecipativo dei tanti magistrati aspiranti alla progressione, sottratti così facendo necessariamente al lavoro giudiziario, e le difficoltà della resa di giustizia, già così afflitta dalla massa di lavoro e dai tantissimi ritardi. Inoltre, i tempi tecnici necessari per l'espletamento delle procedure consiliari di mobilità saranno inevitabilmente allungati dallo svolgimento delle attività delle commissioni di concorso. Le pesanti ricadute sulla mobilità ordinaria dei magistrati, quindi, comprometteranno ulteriormente la qualità della risposta alla domanda di giustizia dei cittadini a causa del prolungamento della scopertura degli uffici giudiziari. Né sarà possibile, per la verità, rispettare in concreto il termine di un anno che la riforma Castelli prevede per la pubblicazione dei posti di secondo grado e di legittimità. di legittimità. Non propongo slittamenti automatici nella progressione in carriera per semplice anzianità, tant'è vero che ho espresso la mia contrarietà al sistema dei ruoli aperti. Vorrei - se consentito dal processo parlamentare - soltanto realizzare qualcosa di ben più energico nel sistema di progressione, cioè un severo controllo quadriennale che non incida sulla resa di giustizia, come ho detto, che non distolga i giudici dal proprio lavoro e che riguardi tutti i magistrati, sia quelli non ancora in condizione di aspirare a funzioni superiori sia quelli che preferiscono curare il difficile compito del primo grado. Comunque, essendo il sistema che propongo fondato sulla raccolta periodica di dati «a futura memoria», ci si pone, così facendo, al riparo - tale è stata un'altra obiezione - da favoritismi correntizi legati di volta in volta all'occasione della promozione. Anche gli incarichi direttivi ricevono notevoli contraccolpi a causa dei limiti di età previsti per le nomine, che determinano una forbice di nove anni tra il momento ultimo di legittimazione all'incarico e la data di cessazione dal servizio, che suscita forte demotivazione ed indurrà i migliori a pensionarsi, come in realtà già sta accadendo. Tuttavia, le conseguenze più gravi si stanno verificando nel nuovo sistema disciplinare e si moltiplicheranno in via esponenziale di mese in mese. Infatti, l'aver introdotto l'obbligatorietà dell'azione e il dovere dei capi di fare rapportoper qualunque lagnanza o esposto che possa profilare un illecito sta intasando, ad oggi, la procura generale della Cassazione, come ha comunicato già da tempo il procuratore generale in una nota a me inviata in data 22 giugno, con la conseguenza di impantanare, a sua volta, la sezione disciplinare e di destinare alla prescrizione (il che è peggio), che la riforma ha ridotto ad un solo anno, anche illeciti che viceversa meriterebbero un'energica sanzione. presidente del CSM, sempre dialogando dal punto di vista istituzionale con il Parlamento, ha pure sottolineato che quel delegato del Ministro, che sarebbe una contrarietà rispetto ad un atto di parità, introdotto dalla riforma Castelli e posto accanto alla pubblica accusa nel procedimento disciplinare, sta suscitando eccezioni di incostituzionalità per evidenti disparità traun'accusa binomica o binaria e una singola difesa; il che porterà ad un ulteriore blocco dell'intero sistema disciplinare. Qui io propongo invece di mantenere l'obbligatorietà dell'azione - come vedete, non è la controriforma - senza però che essa si traduca in una sorta di paralizzante automatismo, prevedendo inoltre un potere di archiviazione da parte della procura generale, in modo da filtrare quanto di inutile le perviene, per poi passare alla sezione del CSM quanto merita un'effettiva trattazione. Poche parole sulle procure della Repubblica. Ho chiaramente detto che condivido l'unitarietà dell'ufficio, l'esigenza di ricondurre i poteri di indirizzo al procuratore e la conferma di una sua ben precisa rappresentatività esterna anche nei rapporti con gli organi di informazione. Ma l'eccesso di verticismo tipico del decreto legislativo n. 109 del 2006 sta deresponsabilizzando i sostituti, come sta accadendo in vari uffici, tanto che il Consiglio è costretto ad intervenire con una circolare del 5 luglio 2006 nel tentativo di dirimere i numerosi contrasti già sorti tra dirigenti e sostituti su singoli aspetti delle nuove norme; insomma, si sta verificando un graduale disimpegno di numerosi sostituti che cominciano a identificare il proprio *status* professionale nella semplice esecuzione delle disposizioni del capo. Vengo al periodo transitorio, e con questo spero di rassicurare il senatore D'Onofrio. Ho proposto un regime transitorio che ridà efficacia alla legislazione precedente, cioè a quella disciplina che non è l'ordinamento del 1941, ma una normativa completamente modificata dai vari interventi e norme successive alla Costituzione. Perché è necessario il periodo di sospensione? Per due motivi fondamentali, a mio parere: innanzitutto, per evitare gli effetti perversi di cui ho parlato e, in secondo luogo, per avere il tempo di approvare le modifiche, sempre con il concorso - mi auguro - della maggioranza e dell'opposizione. Voglio infine anche rassicurare quanti hanno prospettato il pericolo di una ipocrisia istituzionale insita nella sospensione, che diventando permanente farebbe rivivere all'infinito il vecchio sistema.

la congruità del tempo, cioè, nel quale lavorare e costruire questa diversa organizzazione della giustizia nel nostro Paese. Prendo atto delle disponibilità, che pure sono emerse, a confrontarsi serenamente per lavorare insieme agli aggiustamenti da apportare. A mia volta, confermo la disponibilità, purché le prospettive risultino chiare e precise, in linea con i princìpi della Costituzione; siano soprattutto rivolte a non pregiudicare quel servizio giudiziario

un intero corpo dello Stato chiamato ad operare in autonomia e indipendenza a difesa della legalità e che ha avuto anche - non lo dimentichiamo - le sue vittime nell'adempimento dei doveri di ufficio, vittime alle quali va comunque e sempre il commosso ricordo del Parlamento. Presidente, onorevoli colleghi, la mia volontà è ferma nell'idea di operare una costruzione comune e poiché mi è parso di intendere che ci fosse questa analoga volontà da parte di altre componenti dell'Aula, le chiedo, se possibile, una sospensione di un'ora, in modo tale da verificare se esistono queste condizioni; viceversa, nella libera dialettica democratica del Parlamento, ognuno vada avanti. Spero che non sia così e si possa trovare la possibilità di un riscontro effettivo di una volontà comune perché la giustizia in materia istituzionale e ogni fatto istituzionale hanno bisogno di essere confortati dal calore e dalla caloria energetica della maggioranza e dell'opposizione.

Presidente, per motivi regolamentari non sono potuto intervenire durante l'intervento del relatore Salvi e nemmeno durante l'intervento del ministro Mastella,

ho capito quasi nulla di quello che ha detto il senatore Salvi - non ho sentito - e mi è sembrato di percepire che il ministro Mastella abbia avanzato una proposta, verso la fine del suo intervento, della quale, però, non ho udito i termini. Se cortesemente volesse riproporla, con l'Aula che osserva un po' più di silenzio, magari potremmo anche capirci.

Ho sempre la preoccupazione di non interrompere troppo il relatore, chi parla. Resta il fatto che il livello di brusìo e di mormorio è inaccettabile. Visto che giustamente viene rilevato formalmente, mi adopererò perché questa abitudine non dico venga abolita - non sono così ottimista - ma drasticamente ridotta. Su questo piano mi sento realmente impegnato. Ministro Mastella, mi pare che il senatore Castelli le abbia chiesto se vuole ritornare sul punto finale del suo intervento. Se lei lo ritiene, signor Ministro, ha la parola.

di un'ora, laddove ci fossero condizioni di disponibilità, accertate con il mio orecchio, nonostante il brusìo, nelle fasi precedenti la discussione generale.

migliorato; tuttavia, generalmente ci sento benissimo. Il brusìo, negli ultimi undici anni in cui ho frequentato quest'Aula, c'è sempre stato. Posto che questa settimana si discuterà anche il bilancio interno del Senato, le chiedo, signor Presidente, di riconsiderare e di far riconsiderare ai tecnici del Senato il sistema di funzionamento dei microfoni che, al contrario, fin quando i nostri microfoni sono stati pezzi di ottone piuttosto antiquati, ha funzionato perfettamente. Il brusìo c'è, ma l'impianto forse deve essere rivisto.

Mi associo a quanto affermato dal senatore Caruso. Ritengo che, almeno per quanto riguarda il nostro Gruppo, la proposta del Ministro sia assolutamente degna di attenzione. Si tratta di capire in quali termini formali utilizzare la sospensione. Torniamo in Commissione? Facciamo delle riunioni informali? Cosa facciamo? PRESIDENTE. Senatore Castelli, se ho compreso bene lo spirito, forse il Ministro - che può chiarire meglio

segnalando alcune perplessità su questo percorso, che ritengo estremamente asfittico ed accidentato su un tema di fondo. Abbiamo sollevato un problema una netta contrarietà alla sospensione dell'efficacia di una riforma per due terzi entrata in vigore, ed una disponibilità, insieme ad altri partiti dell'opposizione, ad esaminare eventuali proposte di modifica di una legge di impianto, quale è la riforma del centro-destra.

colleghi, il rappresentante del Governo e i Capigruppo chiedono di prolungare di mezz'ora il loro incontro. Sospendo pertanto la seduta fino

di un confronto positivo. Ora, sia da parte dei Capigruppo, sia da parte del Governo, si comunica che il lavoro sta andando avanti positivamente. Naturalmente i risultati si vedranno, se ci sono.